L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia.

assurta agli onori delle cronache nazionali in ragione di una sterile polemica (sono parole del Ministro). Noi, ci permetta, Ministro, non riteniamo tale questa vicenda, perché pensiamo si tratti di un caso di vera e propria discriminazione. I fatti sono molto chiari: il Comune di Lodi adotta una delibera che modifica il regolamento comunale e stabilisce, cito testualmente, che «Ai fini dell'accoglimento della domanda» per l'accesso ai servizi scolastici - stiamo parlando, ad dello scuolabus - «i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre - anche in caso di assenza di redditi o beni immobili o mobili registrati - la certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato esterno corredata di traduzione in italiano legalizzata dall'Autorità consolare italiana che ne attesti la conformità». Già questo ci fa capire come la richiesta formulata sia assurda; una complicazione formulata nei confronti di una categoria ben precisa di persone, a cui se ne aggiunge un'altra, contenuta in una delibera successiva,

Le persone cioè provenienti dall'Afghanistan, dalla Libia, dallo Yemen e dalla Siria, verrebbero esonerate da questa complicazione in più. È come dire, signor Ministro, che quelli che vengono dall'Iraq, dal Sud Sudan, da Haiti e dalla Somalia siano invece nelle condizioni di poter produrre una documentazione che, come lei si rende

dei bambini che dovrebbero invece frequentare gli stessi spazi e usufruire degli stessi servizi esattamente di tutti gli altri. Siamo pertanto a chiederle come ha intenzione di sanare definitivamente una situazione che noi riteniamo inaccettabile.

Presidente, rispondo all'interrogazione evidenziando preliminarmente che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha una specifica e diretta competenza sul servizio di mensa scolastica che, come noto, fa capo agli enti locali, che provvedono all'affidamento dei relativi appalti e stabiliscono in totale autonomia le tariffe da applicare. Ciò non significa che il Ministero sia indifferente al modo in cui viene assicurato dagli enti locali il servizio di mensa nelle scuole, in considerazione del fatto che anche quello del pasto costituisce per le alunne e gli alunni un momento di arricchimento educativo e di condivisione. Quanto allo specifico quesito postomi, fornisco alcuni chiarimenti condivisi con il Ministero dell'interno. (ISEE) è, come noto, lo strumento di valutazione attraverso il quale viene determinata la situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. L'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, stabilisce che l'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello DSU, ovverosia la dichiarazione unica sostitutiva in riferimento al nucleo familiare, prodotta ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Il predetto testo unico, all'articolo 3, prevede che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani o nel caso in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. Al di fuori dei citati casi, gli stati, le qualità personali e i fatti devono essere documentati mediante la produzione di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana. Pertanto, la delibera del Comune di Lodi si è limitata da applicare, con riferimento alla situazione reddituale o economica, la disciplina vigente, prevedendo peraltro delle eccezioni in favore di cittadini extracomunitari aventi lo *status* di rifugiato politico, nonché di quelli appartenenti a Paesi in cui è oggettivamente impossibile acquisire la documentazione

guida volte a facilitare ulteriormente i cittadini extracomunitari nella dimostrazione del possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni economiche per l'accesso dei propri figli al servizio di mensa scolastica. Concludo con l'invito a non strumentalizzare episodi isolati, in quanto si corre solo il rischio di alimentare il contrasto sociale, perdendo invece di vista l'importanza di azioni di sistema, come quelle poste in essere in pochi mesi da questo Governo, che ha predisposto significative misure per i giovani, per le famiglie e per il contrasto alla povertà.

la facoltà di entrare in questa vicenda, che non è quello di competenza. Noi, per la verità, avevamo rivolto questa interrogazione al ministro Salvini, ma poco importa che abbia risposto lei, perché è membro di

questa operazione. State facendo un'operazione tutta politica sulla pelle dei più deboli. In questo caso sono deboli quei soggetti, perché vengono da altri Paesi, da condizioni complicate e ho fatto riferimento all'elenco di Paesi che sarebbero all'elenco di Paesi che sarebbero esonerati da quest'obbligo proprio per dire che stiamo parlando, comunque, di vicende molto complicate. Tuttavia, sono deboli quei soggetti perché sono innanzitutto dei bambini

con la spiegazione burocratica che abbiamo sentito poco fa: quello che è successo a Lodi è un fatto grave di discriminazione. Un Ministro dell'istruzione deve porsi la finalità di garantire a tutte le bambine e a tutti i bambini di questo Paese il diritto-dovere di andare a scuola e di accedere a tutti

qualsiasi amministrazione, di qualunque colore politico, quelle bambine e quei bambini vadano a scuola e assolvano al loro diritto-dovere. Questo va al di là delle competenze, perché è una competenza che riguarda

qualcuno ha raccontato a quei bambini che un certo bambino, all'ora della mensa, non poteva più stare con loro. Il fatto che una comunità si sia mossa, si sia attivata, abbia raccolto dei fondi, abbia avuto la capacità di reagire, che è un fatto positivo, non può essere la risposta di uno Stato civile, di uno Stato europeo, di uno Stato del G7 di fronte a un tema come questo. Non può essere questo. Voi dovete dare un segnale che sia esattamente il contrario di ciò che è accaduto in queste settimane, quando un'amministrazione comunale, in maniera ideologica, ha utilizzato vigliaccamente un cavillo burocratico per fare della discriminazione, non avendo neanche il coraggio

genitori, che provenivano dai Paesi più vari (ma molti erano italiani) e magari non pagavano quel servizio. Non ho mai pensato - e nessuno di noi ha mai pensato - di non fornire il servizio ai bambini. Ecco, di fronte ad un'amministrazione che si comporta così, uno Stato, un Ministero interviene subito e fa capire a tutte le amministrazioni che nessuno può permettersi di fare questo in Italia. Invece, questo Governo ha dato una copertura politica a quel comportamento e ha creato le condizioni perché anche altre amministrazioni lo facciano. Io le chiedo di invertire la rotta e di dirci che cosa intende fare e anche quali sono quei progetti per i giovani che adesso lei ha annunciato ma che noi non abbiamo ancora individuato nell'azione di governo. Presidente, rispondo all'interrogazione ribadendo quanto poc'anzi evidenziato nella risposta ad analoga interrogazione, ovvero che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha una specifica diretta competenza sul servizio di mensa scolastica che, com'è noto, fa capo ai Comuni, il che non significa che il Ministero sia indifferente al tema, in quanto disporre di mense scolastiche vuol dire poter offrire il tempo pieno a scuola e così sostenere le famiglie, dando un'opportunità di scelta più articolata ai fini educativi. Vengo adesso a quanto lei ha chiesto. Il predetto Dipartimento ha pertanto concluso che nel caso verificatosi a Lodi non è stato violato alcun diritto, in quanto l'accesso a scuola e all'insegnamento primario è stato garantito a tutti gli alunni a prescindere dalla nazionalità. Il medesimo Dipartimento ha altresì escluso che vi sia stata violazione delle direttive europee in tema di non discriminazione sulla base della nazionalità e dello *status* di immigrazione, in quanto la delibera del Comune di Lodi del Comune di Lodi «È finalizzata a fotografare la situazione reddituale e patrimoniale dei cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, proprio al fine di non creare discriminazioni nell'accesso dei servizi accessori della scuola». Per quanto riguarda, invece, la richiesta relativa a quali iniziative intenda intraprendere, nel ribadire che la normativa rimette all'autonomia degli enti locali la gestione del servizio di mensa, che deve essere organizzato e modulato secondo la reale necessità dei territori in ragione della specificità del contesto socio-economico locale, non posso che sottolineare come non si debbano generalizzare casi isolati, le cui conseguenze sono state ingigantite, atteso che, per per come riferito dal competente ufficio scolastico di Lodi, gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa sono in numero limitato ed in linea con gli anni passati. La scuola, la più importante istituzione del nostro Paese, che ha il delicatissimo compito di formare le nuove generazioni, non merita, come purtroppo spesso accade, di essere coinvolta in sterili strumentalizzazioni e polemiche. *(Applausi dai Gruppi

perché lei qui aveva l'opportunità di parlare da Ministro dell'istruzione e da uomo di scuola, quale lei è, e le parole che lei ha qui pronunciato, nella risposta precedente e in quella riguardante la nostra interrogazione, non sono parole da uomo di scuola e tantomeno da Ministro della pubblica istruzione. Lo dico perché lei ha rilasciato tante interviste, da settembre, ha cercato di barcamenarsi tra quelli che erano i diritti dei bambini e i doveri dei genitori, che nessuno ha mai messo in discussione, perché quegli stessi genitori vogliono pagare, chiedono solo di essere messi nella condizione di dimostrare quello che hanno e quello che non hanno, per poter pagare il giusto, né più, né meno. Si tratta, quindi, di un discorso di giustizia. Ma alla fine di tutto questo, Ministro, la sua voce doveva sentirsi, perché quelli che hanno pagato il conto non sono stati neanche i genitori, ma sono stati quei bambini che hanno pagato il conto della separazione e della discriminazione rispetto ai loro compagni di classe e un Ministro dell'istruzione, a prescindere dal fatto che questa non sia squisitamente la competenza tecnica del suo Ministero, su questo interviene e lo dice ad alta voce. Dice che quel fatto che è successo a Lodi e che purtroppo sta cominciando a dilagare in altri Comuni dell'*hinterland* milanese, è un fatto indegno. Forse interessa a tutti voi mantenere sempre quel certo clima di tensione che piace così tanto anche al Ministro che le siede a fianco, che si ricorda di essere padre, ma probabilmente non nutre lo stesso affetto nei confronti dei bambini che la pelle bianca non ce l'hanno. Lei che è uomo di scuola,

detto, quando il ministro Salvini ha preso le difese della sindaca di Lodi e ha detto che andava bene così? Ministro, purtroppo al grido di «prima gli italiani», ci vanno di mezzo sempre i più deboli. Lei ha giurato sulla Costituzione: l'unico *slogan*, l'unico elemento che lei deve tenere in considerazione è «prima i bambini». Questo le viene chiesto.

nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2018-2019. Ebbene, solo 25.105 (ovvero il 43,8 per cento) sono andate a buon fine, ben sei cattedre su 10 sono rimaste vacanti e il dramma è sul sostegno, dove su 13.329 posti sono stati assunti solo 1.682 insegnanti, il 12,6 per cento. Il sistema di reclutamento, quindi, va aggiornato, perché in questo modo probabilmente fa acqua. La graduatoria, ormai ferma al 2016, è in esaurimento e dei tre concorsi previsti per quest'anno solo uno è in corso. All'inizio dell'anno scolastico, è proprio al Nord, ahimè, che è stato assegnato il minor numero di cattedre, quasi 13.000 su oltre 34.000. Un po' meglio va al Centro (41 per cento) e al Sud (63 per cento). Nella mia Regione, la Lombardia, non c'è solo una carenza di insegnanti, ma su un numero totale di 1.142 scuole mancano qualcosa come 329 dirigenti scolastici e sono quasi 500

675 unità, suddivise tra i vari ambiti territoriali provinciali. Le presenze effettive risultano invece essere meno della metà. Nell'ufficio scolastico territoriale della mia Provincia, quindi della Provincia di Bergamo, su 72 presenze previste solo 22 risultano effettive e questo è un vero e proprio grido di aiuto, perché, signor Ministro, il personale amministrativo degli uffici scolastici territoriali della Lombardia si trova veramente a fronteggiare grandi difficoltà organizzative per cercare di garantire il corretto proseguimento dell'anno scolastico, attraverso un'intensificazione dell'attività lavorativa - alla bergamasca direi - arginando encomiabilmente il malumore di studenti e genitori al ripetersi di situazioni di disagio che portano sempre più spesso alla riduzione quindi che resta necessario indire nuovi concorsi per i docenti di ruolo e soprattutto per quelli di sostegno, per non dover mettere nuovamente gli uffici scolastici regionali in condizioni di compiere i miracoli in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, è altrettanto urgente adottare iniziative al fine di risolvere la situazione di carenza di organico in cui versano i suddetti uffici. Signor Ministro, lei non è solo un uomo di scuola, ma è stato anche dirigente dell'ufficio scolastico regionale Lombardia nell'ambito territoriale di Milano, per questo mi rivolgo a lei in maniera particolarmente accorata. Questo mi conforta, perché la sua esperienza e l'amore per la scuola saranno effettivamente elementi determinanti

delle istituzioni scolastiche nella loro attività quotidiana; sono altrettanto consapevole del fatto che, ormai da anni, gli uffici scolastici soffrono di una grave carenza di organico che interessa tutte le Regioni d'Italia e che è stata determinata dagli stringenti vincoli assunzionali imposti, nel recente passato, a tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresa quella scolastica. A queste gravi carenze ha fatto fronte il personale amministrativo in servizio. Grazie all'encomiabile impegno di tale personale è stato possibile ovviare alle difficoltà organizzative e garantire il corretto inizio e il regolare svolgimento dell'attività scolastica nel corso di tutti questi anni; a tale personale, come a tutto il personale della scuola, va il mio sentito ringraziamento. Le difficoltà in cui versano gli uffici scolastici territoriali saranno, almeno in parte, attenuate con il reclutamento di 253 funzionari di area III, con competenze di natura amministrativa, giuridica e contabile, le cui procedure di assunzione sono in corso di espletamento e che saranno presto destinati alla sede centrale e alle sedi periferiche dell'Amministrazione. La prova preselettiva del concorso si è svolta nei giorni 27 e 28 settembre e in data 3 ottobre, è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta. Assicuro che vigilerò perché l'*iter* concorsuale si concluda nel più breve tempo possibile. Aggiungo che il piano di programmazione triennale delle assunzioni, che ho trasmesso il 25 settembre scorso al Dipartimento della funzione pubblica, prevede, oltre all'assunzione dei vincitori del concorso al quale ho fatto riferimento poc'anzi, di bandire una nuova procedura concorsuale per reclutare altri 95 funzionari e di assumere gli idonei di vari concorsi, anche banditi da altre amministrazioni. Quest'ultima iniziativa consentirà di assumere rapidamente il personale e di destinarlo alle sedi che si trovano in situazione di maggiore sofferenza. Proprio in tale ottica e nella consapevolezza delle particolari difficoltà in cui versano gli uffici scolastici territoriali delle Regioni settentrionali del Paese, in particolare quelli della Lombardia, ho, da poco, firmato una direttiva che dà precise indicazioni alla competente direzione del Ministero su come ripartire il contingente di personale da assumere, dando assoluta priorità proprio a tali uffici.

ancora concorsi *ad hoc* non ne vediamo. Nell'attesa, comunque, che la situazione del personale scolastico si sblocchi, ritorno soltanto per un momento sulla che sono veramente prossimi al collasso, con l'aggravante che, a causa del blocco del *turnover*, i pochi lavoratori più giovani superano i quarant'anni di età, mentre gli altri si attestano in media sui cinquantotto anni. Se va in pensione l'unico lavoratore adibito a uno dei servizi dell'ufficio scolastico territoriale, quello chiude perché manca il sostituto: è il caso,

signor Ministro: noi saremo con lei, ovviamente, in tutto quello che si potrà fare. È una grande responsabilità, perché garantire il diritto allo studio, come da Costituzione, è sacrosanto.

Premesso che: nei giorni scorsi un furgone della gendarmeria francese è stato avvistato dalla Polizia italiana nei pressi di Clavière, Comune dell'Alta Val di Susa, nella città metropolitana di Torino, mentre faceva scendere alcune persone, molto probabilmente dei migranti di origine africana, in una zona boschiva poco prima del *tunnel* di Cesana Torinese, adiacente al confine di Stato; dopo aver compiuto tale operazione, il furgone è poi rientrato in territorio francese; la Polizia italiana ha provveduto ad annotare la targa e ad avviare una serie di indagini sui fatti; nelle registrazioni in possesso della Digos, si scorge il furgone, mentre farebbe scendere i presunti migranti, i quali si sono poi incamminati nel bosco facendo perdere le loro tracce; la Digos ha trasmesso le immagini alla Procura di Torino, che ha prontamente aperto un fascicolo; qualora i fatti fossero confermati, si tratterebbe di un precedente molto grave, in quanto, alla luce degli accordi internazionali vigenti, in casi del genere l'Autorità straniera è tenuta ad avvertire il commissariato di Polizia o la stazione dei Carabinieri di zona; non si può escludere che vi siano stati tentativi di condurre in territorio italiano anche migranti minorenni, secondo quanto denunciato da numerose organizzazioni e da alcuni sindaci dei comuni

secondo quanto riportato dai principali quotidiani, la Prefettura della regione francese Hautes-Alpes avrebbe parlato a tal proposito di un "errore" commesso da gendarmi a motivo del fatto che gli stessi erano in servizio da pochissimi giorni nella regione e non conoscevano bene il la Prefettura avrebbe poi precisato che, nell'ambito di una missione di rimpatrio di stranieri irregolari, un veicolo della gendarmeria francese avrebbe attraversato il confine franco-italiano in direzione di Clavière,

è vero, senatore: le autorità francesi infrangono la legge, ripetutamente. Nella mattinata del 13 ottobre - è ormai evidente - il personale della Digos ha notato nel Comune di Claviere un furgone della gendarmerie, dal quale scendevano due giovani stranieri che si avviavano verso i boschi. L'episodio ha dato origine all'apertura, da parte della procura della Repubblica di Torino, di un'indagine per il reato di trasporto di stranieri nel territorio dello Stato. Le autorità, di fronte alla richiesta di una spiegazione, hanno parlato di un deplorevole errore, annunciando una indagine interna, ma è evidente che abbandonare immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore o un incidente. Quanto successo a Claviere è un fatto evidentemente grave, anche perché non si tratta di un fatto isolato: è di questi minuti la denuncia della Croce Rossa di Ventimiglia dell'allontanamento di due minorenni spacciati per maggiorenni, addirittura, dalle autorità francesi al confine con l'Italia, e sono numerose le altre testimonianze di illegalità commesse dalle autorità francesi, alla faccia di qualsiasi accordo o trattato internazionale. Cosa stiamo facendo? Ovviamente abbiamo intensificato i controlli; abbiamo mandato pattuglie della Polizia di Stato; chiediamo alle autorità francesi di conoscere nomi, cognomi, età e nazionalità di coloro che sono stati respinti, ricordando i 50.000 respinti dal 1° gennaio dell'anno scorso ai confini fra Francia e Italia e, soprattutto, non accettiamo lezioni, non accettiamo lezioni, né dai francesi, né dalla sinistra italiana perché rispettiamo le regole. Abbiamo accolto 700.000 persone negli ultimi anni, ma quando è troppo è troppo. Abbiamo semplicemente ripristinato i controlli alle frontiere, in attesa che l'Europa muova un dito. L'Europa è molto pronta a mandare letterine all'Italia sulle manovre economiche e molto distratta quando si espellono bambini spacciandoli per maggiorenni, che è una bestialità che va ben oltre quanto ho sentito prima. *(Applausi In attesa della letterina che da Bruxelles arriverà a Parigi, facciamo per conto nostro; verifichiamo che si rispettino le leggi e, intanto, il dato che vi do aggiornato a oggi grazie a una politica seria i 111.000 sbarchi dell'anno scorso quest'anno sono fermi a 21.000 e il miliardo di euro risparmiato servirà a mettere meno soldi in tasca alle coop e ai finti profughi e a garantire 10.000 uomini delle Forze dell'ordine per la sicurezza del nostro Paese.

una condizione ancora peggiore la vivono i lavoratori del comparto (agenti della polizia penitenziaria, dell'amministrazione della giustizia, sanitari e volontari che prestano servizio). Bastano pochi dati per rendersene conto. Al mese scorso i detenuti nei penitenziari di tutta Italia sono quasi 60.000. A giugno erano 58.000, in continuo aumento, a fronte di una capienza regolamentare di poco più di 50.000. Al contrario, l'organico della polizia penitenziaria è di soli 35.000 unità rispetto alle 41.000 previste, circa il 15

La traduzione pratica di questi numeri è che gli agenti sono costretti a turni massacranti e in numero inferiore alle condizioni minime di sicurezza. Solo per fare un esempio, nel carcere di Teramo, che ho visitato, 130 effettivi coprono il lavoro di 220 unità, con 150 reclusi in sovrannumero. Hanno accumulato 16.000 giorni di ferie non godute, 45.000 ore di straordinario e la regola è lo svolgimento di turni massacranti,

si registrano percentuali di vacanza che arrivano all'83 per cento per i commissari e scendono, comunque, al 16 per cento per agenti e assistenti. Le condizioni di sicurezza in cui lavorano questi agenti, spesso oggetto di frequenti aggressioni, sono aggravate dalla presenza tra gli stranieri di migliaia di detenuti islamici sensibili alla radicalizzazione violenta e ancora più precarie sono rese dall'introduzione della cosiddetta vigilanza dinamica. Si tratta di una bella invenzione che prevede la libera circolazione di detenuti negli spazi comuni

e che sono oggetto delle nostre domande (impegni che, peraltro, condividiamo nel merito). Chiediamo al Governo di stanziare i fondi per assumere il personale e completare la pianta organica. Invece di distribuire reddito di cittadinanza, usiamo meglio le risorse e creiamo lavoro vero.

di tornare indietro rispetto alla cosiddetta riforma Orlando e soprattutto alla vigilanza dinamica; di sviluppare il ricorso, finora marginale, all'impiego dei detenuti per lo svolgimento di lavori di utilità sociale,

la rieducazione dei detenuti e la messa in sicurezza delle condizioni in cui lavorano gli agenti di polizia penitenziaria, che svolgono un lavoro importantissimo non solo non solo per la sorveglianza in senso stretto dei detenuti, ma anche in termini di prevenzione. Infatti, i detenuti che rientrano nella società devono aver fatto un percorso di rieducazione; se lo avranno fatto, non torneranno a delinquere. del monitoraggio importante che la polizia penitenziaria svolge in termini di prevenzione del terrorismo e della mafia. Con particolare riferimento alla carenza di organico - è un dato tristemente diffuso su tutto il territorio nazionale - lo Stato si attesta su un tasso di scopertura complessivo pari al 9,9

del Corpo di polizia penitenziaria nominati al termine del relativo corso di formazione *in itinere*, nonché l'attivazione delle procedure per il concorso interno per complessivi 2.851 posti per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo maschile e femminile. In ogni caso, richiamo l'investimento di 500 milioni di euro per il personale di sicurezza, in cui rientra anche il personale della polizia penitenziaria.

60.000 posti, sono già in atto procedimenti avviati dal Piano carceri, attualmente curati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per nuovi istituti e padiglioni, per circa 3.800 nuovi posti regolamentari.

Ora, ci siamo già attivati per sbloccare i soldi che già c'erano e venivano lasciati lì; non solo: al Ministero c'è un gruppo di lavoro che, in versione *task force*, sta cercando di lavorare per valutare per valutare la possibilità di riconvertire in tempi urgentissimi alcune caserme militari dismesse, al fine di provvedere all'emergenza dell'edilizia penitenziaria, non solo in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche di nuove carceri, là dove necessario. Per quanto riguarda l'invito a valutare la possibilità di far espiare la pena ai detenuti stranieri nei loro Paesi di provenienza, sottolineo che c'è un impegno non solo da parte del Ministero della giustizia ma anche del Ministero dell'interno a intrattenere il maggior numero possibile di rapporti diplomatici con i Paesi maggiormente

com'è noto, è stata bloccata nella parte in cui configurava l'ennesimo svuotacarceri, che poi avrebbe comportato anche problemi per la sicurezza degli agenti di polizia penitenziaria. È rimasta invece la parte di quella riforma che va incontro alle esigenze di tutti, soprattutto

Non ci ha dato rassicurazioni sulla vigilanza dinamica; anzi, mi sembra di capire che, quando difende un parte della riforma Orlando entrata in vigore per far stare meglio dentro alle carceri forse si riferisce proprio a questo, ma casualmente non ne ha parlato. Sono anche poco soddisfatto del fatto che consideriate il taser un'arma pericolosa, con la conseguenza che le persone che subiscono aggressioni dentro alle carceri debbano difendersi a mani nude, come oggi accade, e in grave inferiorità numerica, anche a causa delle deficienze di personale.

buonista di coloro che pensano che stare dalla parte dei più deboli significhi invertire il senso comune delle cose, al punto da pensare più a quanto siano maltrattati i poveri detenuti che alle condizioni concrete e reali di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria. Si tratta peraltro della stessa subcultura che porta il vice della sindaca Raggi a incontrare e difendere gli occupanti abusivi, mentre il Ministro dell'interno tenta di dar vita a una stagione di sgomberi e demolizioni, che attendiamo di vedere con ansia, ma della quale finora non abbiamo ancora visto alcun atto pratico. Naturalmente diamo tempo al tempo:

Signor Presidente, signor Ministro, premesso che violenza contro le donne è ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica, per le donne, incluse minacce, coercizione, privazione arbitraria della libertà. Premesso ancora che, come dimostrato dai dati statistici ufficiali e dalle numerose richieste di aiuto delle vittime di violenza domestica, *stalking* o abusi sessuali presso gli appositi centri di ascolto dislocati sul territorio nazionale, si tratta di un fenomeno in costante crescita. A questo dev'essere poi aggiunto,

o minorenni per paura delle conseguenze o perché si sentono ingiustamente colpevoli di una simile aggressione;

quali iniziative ha intenzione di intraprendere volte al contrasto di questo problema che sta assumendo le vesti di una vera e propria piaga sociale.

la senatrice interrogante, premessa la costante crescita delle vittime di violenza domestica, *stalking* o abusi sessuali, chiede quali iniziative il Ministro intenda assumere, anche sul piano normativo, per contrastare il fenomeno della violenza di genere. Partiamo da un presupposto: la piaga della violenza di genere non è soltanto una piaga sociale, ma è una piaga culturale, una piaga tragica che deve vedere tutte le forze politiche - come sicuramente sicuramente vedrà - impegnate in un contrasto che deve essere netto e deve - lo ribadisco - agire in termini di prevenzione prima di tutto culturale. Nella scorsa legislatura è stata ratificata la Convenzione di Istanbul,

giustissimo l'inasprimento delle pene, ma sappiamo tutti che esso non ha una funzione deterrente nei confronti di questo tipo di reati. Uno che vuole pagare una mazzetta nutre nella sua mente il pensiero e si pone il dubbio su cosa pagherà in termini di carcere nel momento in cui verrà beccato con la mazzetta; ma uno che sta esercitando una violenza nei confronti di una donna non si sta ponendo il problema delle pene cui andrà incontro successivamente. Ciò impone allo Stato di agire in prevenzione. Da questo punto di vista oggi è stato presentato al Ministero della giustizia il disegno di legge recante modifiche al codice di procedura penale e disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. È il cosiddetto codice rosso: si tratta di interventi che provano ad agire in prevenzione. Quando cioè una donna decide con grande fatica, attraverso un percorso di coraggio che non bisogna dare per scontato, di rivolgersi allo Stato magari per denunciare la violenza domestica che sta subendo, in quel momento lo Stato deve attivarsi con immediatezza, come accade al Pronto soccorso di fronte a un caso grave. Per cui questo disegno di legge, che possiamo riassumere come «codice rosso», prevede che l'agente o il pubblico ufficiale che riceve la denuncia debba immediatamente darne comunicazione, senza possibilità di discrezionalità sulla valutazione

atti di indagine, la polizia deve dare una preferenza ed agire con immediatezza; e dopo che ha compiuto le indagini, sempre con immediatezza, deve informare il pubblico ministero. Inoltre, è prevista - ed è per questo che c'è il concerto con il ministro Giulia Bongiorno, che ha fortemente voluto questo provvedimento e che ringrazio qui pubblicamente per la splendida collaborazione e interlocuzione

che avranno la possibilità di interloquire con la denunciante. Tutti questi aspetti sono fondamentali, perché noi diamo per scontato che in un Pronto soccorso ci si vada quando qualcuno ha

di richiesta di aiuto, tenderle la mano e accompagnarla in un percorso di protezione, che è qualificato non solo nei tempi di risposta ma anche nella qualità della risposta e del sostegno. Il Governo è fortemente impegnato sulla protezione delle donne donne e comunque contro la violenza di genere. Abbiamo diversi tavoli attualmente attivi: il primo alla Presidenza del Consiglio riguardante il Piano nazionale antiviolenza coordinato dal sottosegretario Vincenzo Spadafora, al quale il nostro Ministero partecipa attivamente, e il secondo riguardante la tutela delle vittime di reato in genere. Stiamo lavorando, infine, al Fondo delle vittime dei reati internazionali violenti con il fine di aumentare l'ammontare degli indennizzi da riconoscere alle vittime ed eliminare alcuni paletti normativi che ne precludono l'accesso. Permettetemi di precisare quanto sia importante che la giustizia venga percepita dei nostri cittadini non come un'entità che si incrocia quando le cose sono andate male e quando non c'è più la possibilità di tornare indietro; mi piace pensare che i cittadini pensino, immaginino e percepiscano la giustizia italiana come un settore su cui lo Stato investe e che ti viene incontro in una fase di prevenzione quando ancora il reato non è stato commesso. Se questo vale in generale per tutti, vale nei confronti di tutte quelle donne che in Italia subiscono violenze da chi pensa di potersi considerare uomo sfruttando la propria forza fisica, e che invece non può essere considerato nemmeno «persona», non uomo ma nemmeno persona, perché sono gli animali che pensano di poter sopraffare

Signor Presidente, sono molto soddisfatta di quanto appreso dal Ministro, a dimostrazione della sua sensibilità a questa problematica. Confido nel superamento di tali situazioni conflittuali che portano giornalmente ad eventi drammatici cui si assiste quasi impotenti. La ringrazio, signor ministro Bonafede.

maggiormente la vicinanza alla sua famiglia, alle sue amiche, ai suoi amici, ai suoi coetanei di sedici anni. Ma da oggi in poi ognuno di noi deve fare la sua parte per garantire la sicurezza e la libertà delle nostre figlie. *(Applausi agitatissima la sera quando mio figlio non torna. È questo però il mestiere di genitori e dobbiamo garantire loro libertà e benessere sociale ai cittadini e alle cittadine. In particolare, siamo vicini ai cittadini e alle cittadine del quartiere San Lorenzo, strapieno di giovani: è bellissimo andare lì la sera, perché lì i ragazzi e le ragazze si ritrovano. Come dicevo, però, dobbiamo essere vicini ai cittadini e alle cittadine di quel quartiere per risolvere situazioni di degrado

evince che le Forze dell'ordine denunciano una carenza di personale e non ce la fanno a garantire la sicurezza sul territorio. C'è una lettera dell'amministrazione municipale in cui si sollecita l'intervento della prefettura, che è l'organismo deputato a garantire la sicurezza e a risolvere il problema di quel sito. Dico allora di nuovo, da madre,

Signor Presidente, onorevoli senatori, purtroppo mi vedo costretto a segnalare oggi in quest'Aula il ripetersi di incresciosi episodi che vedono coinvolta la mia terra, la Basilicata, dove c'è un Presidente di Regione che ha trascorso quasi novanta giorni agli arresti domiciliari, misura trasformata oggi in divieto di dimora nel capoluogo, Potenza, che poi è la sede del Consiglio regionale e della Giunta. notizia di due giorni fa quella di una nuova inchiesta della magistratura che ha messo sotto indagine l'intera Giunta regionale, e quindi ancora il governatore Pittella, per casi di malasanità e per abuso d'ufficio riguardo alle nomine di alcuni

Ai lucani questo comparto costa ben 1,3 miliardi di euro, quasi la metà dell'intero bilancio regionale. Che cosa produce? Malasanità, migrazione sanitaria, chiusura degli ospedali e avvisi di garanzia alternati ad ordinanze di custodia cautelare. soprattutto, di un'area economica depressa e quindi di un comparto che interviene a consumare, come già detto, quasi la metà del bilancio regionale, provocando quindi dei grandi pericoli per l'insediamento di infiltrazioni mafiose, oltre a favoritismi, clientele, appalti, consulenze, assunzioni e chissà cos'altro. Del rischio dell'insediamento della mafia in Basilicata non parlo io; che ci sia la mafia in Basilicata lo dice il procuratore distrettuale antimafia di Potenza Francesco Curcio. Che in Basilicata l'intreccio tra mafia e politica è ben ingranato e oliato non lo dico io, ma l'ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, il quale nel 2017 parlava di una certa abilità della mafia lucana, rispetto alle altre mafie, a intrecciare rapporti con politici locali e amministratori.

manifestando lo sdegno per un Presidente di Regione che non si dimette a fronte di una grave misura cautelare, mantenendo invece in vita un Consiglio regionale che ancora promuove incarichi, consulenze e chissà quant'altro.

Sembra di stare nei cartoni animati dei «Simpson»; laddove ci sono delle inchieste che coinvolgono tutta la Giunta regionale questa, anziché dimettersi e mostrare una certa dignità al popolo lucano, chiede di andare avanti ancora.

mentre loro chiedono il rinvio delle votazioni, io oggi chiedo invece che si vada subito al voto, che si vada al voto prima della fine dell'anno, magari prima di Natale. Non è una richiesta personale, ma la richiesta di un popolo stanco di essere sfruttato e ostaggio di una una politica totalmente assente.